Onorevoli colleghi, sessantaquattro anni or sono, in questo giorno di gennaio, le truppe russe raggiungevano, nella loro avanzata verso Ovest, il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, abbandonato dai nazisti in fuga. Campo che tanti giovani, tanti di voi ed io stesso abbiamo visitato nel corso degli anni con commozione profonda. L'apertura dei cancelli restituì la libertà alle migliaia di sopravvissuti all'atroce meccanismo dello sterminio, e mostrò a tutto il mondo quanto era accaduto in quei luoghi di dolore, che da anni accoglievano senza sosta convogli di deportati provenienti da tutta l'Europa occupata. A partire da quel giorno, nessuno poté più dire di non sapere o di non aver compreso: la meticolosa determinazione delle truppe liberatrici alleate, nel documentare l'orrore che si trovarono dinanzi, in quello e in tanti altri campi, consegnava alla storia le prove viventi ed i terribili risultati dell'osceno disegno - perseguito con metodo dalla lucida follia omicida dell'ideologia nazista di cancellare il popolo d'Israele, e tanti altri esseri umani, dalla storia e dalla geografia del nostro continente. Per questo la Repubblica italiana riconosce, ormai da nove anni, il 27 gennaio quale «Giorno della Memoria», al fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, l'infamia delle leggi razziali, la persecuzione dei cittadini di religione ebraica e di tutti gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia e la morte nei campi nazisti. Fare memoria significa oggi «considerare che questo è stato», secondo le parole di Primo Levi. Significa interrogarsi sulle ragioni storiche e i meccanismi politici e culturali che permisero al sentimento antisemita, radicato in settori della società tedesca ed europea, di tramutarsi dapprima nel cuore dell'ideologia nazista, e poi in un lucido e determinato disegno di persecuzione e di sterminio, alla cui realizzazione fu destinata ampia parte delle energie militari ed amministrative del regime hitleriano e dei suoi alleati. Significa riconoscere che quell'orrore si sviluppò nel cuore della civiltà europea, dissipando in un istante, insieme alla dignità umana di quanti caddero vittime della persecuzione e dello sterminio, quel patrimonio di principi e di valori che quella medesima civiltà europea aveva faticosamente e coraggiosamente costruito. Significa non stancarsi di denunziare il sentimento antisemita tuttora presente in una parte consistente della nostra società (circa il 12 per cento della popolazione, secondo i più recenti sondaggi), spesso travisato sotto la maschera altrettanto odiosa dell'antisionismo, cioè dell'atteggiamento di chi non riconosce allo Stato di Israele neppure il diritto di esistere. Nel momento in cui, nella politica e nella società, si iniziasse a pensare al diverso da sé come un nemico da abbattere, allora si porrebbero, come scrisse Vittorio Foa nella prefazione all'opera di Primo Levi, le premesse di una catena inesorabile, al cui termine c'è il *lager*. Fare memoria significa anche però onorare il valore di quanti riuscirono, in quei difficili momenti, a rimanere fedeli alla propria natura umana e ad opporsi con coraggio a quell'odioso progetto di morte, adoperandosi, spesso a rischio della propria vita, spesso in un silenzio operoso, per sottrarre anche un solo fratello perseguitato al suo terribile destino. il Memoriale dell'Olocausto di Gerusalemme, dedica alla memoria di costoro, nominati «Giusti tra le nazioni», una distesa di piccole lapidi poste lungo il viale alberato che conduce alla Tenda della rimembranza, dove arde la fiamma perenne che ricorda le vittime della Shoah. In occasione della mia visita al Memoriale, nello scorso settembre, sono rimasto commosso e inorgoglito nel constatare come a molte di quelle lapidi corrisponde il nome di un cittadino italiano. Quelle storie di umanità e coraggio, ricostruite e pubblicate negli ultimi anni a cura della Commissione per il riconoscimento dei Giusti italiani, rappresentano una pagina luminosa della storia del nostro Paese e contribuiscono a riscattare la memoria dolorosa delle leggi razziali. Alla memoria di questi uomini giusti, accanto a quella di quanti patirono nel corpo e nello spirito gli effetti di quella brutale violenza, si rivolge oggi il nostro pensiero commosso e l'invito alle giovani generazioni a conoscere e a non dimenticare. Invito pertanto l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento.

i cancelli di Auschwitz, il più grande campo di concentramento della Germania nazista, venivano abbattuti. Da lì a poco tutti gli altri campi di concentramento sarebbero stati smantellati e la Seconda guerra mondiale avrebbe cancellando nazismo e fascismo e aprendo in Italia e in molti altri Paesi europei la fase democratica. Quello che è accaduto in quei campi però non può, e per fortuna non è stato cancellato. Letestimonianze, i ricordi dei sopravvissuti, i filmati dell'epoca lasciano ancora vivo in noi il dolore per milioni di vite umane spezzate dalla follia, sterminate, umiliate, perseguitate dalla brama criminale della dittatura nazista. Sei milioni di ebrei trucidati, senza dimenticare i rom, i sinti, gli omosessuali, i prigionieri di guerra, i disabili, i malati di mente, i testimoni di Geova, i prigionieri politici e tutte le altre "categorie" sacrificate per giustificare le indegne teorie sulla purezza della razza. La Shoah è una pagina tremenda che il Novecento ci ha lasciato in eredità. Una discesa nell'abisso, un inferno in terra, il progetto genocida di pochi uomini, ma anche di molti testimoni muti, silenziosi, dunque complici. Giornate come queste non sono allora un semplice momento di riflessione fine a se stesso, ma servono a tenere vivo quel ricordo, ad essere monito per tutti noi, ma soprattutto per le giovani generazioni. Ciò che accadde nei campi di concentramento della Germania nazista non solo non deve più ripetersi, ma non deve nemmeno essere oggetto di letture alternative, di strane interpretazioni, di deprecabili emulazioni. Non ci sono «letture altre» ad un dramma come quello dell'Olocausto, alle testimonianze dei pochi reduci, agli incontrovertibili documenti arrivati fino ai giorni nostri. Ilrischio è che a distanza di decenni le popolazioni ebraiche siano ancora minacciate. Il pericolo è tutt'altro che lontano: ci sono *leader* di Nazioni, penso all'iraniano Ahmadinejad, che considerano l'Olocausto «un sogno», e che vorrebbero la distruzione di Israele e la sua cancellazione dalla carta geografica. Allo stesso modo, esistono sacche di antisemitismo e di xenofobia che sono certamente minoritarie ma che non possono essere sottovalutate. In Italia l'antisemitismo non è ancora del tutto sconfitto. Pensiamo a ciò che è successo nel nostro Paese durante la guerra di questi giorni nella striscia di Gaza tra Israele e i miliziani di Hamas. Bandiere con la stella di David bruciate, manifestazioni di aperto antisemitismo nelle piazze, scritte offensive sui muri: c'è chi, a Roma, è arrivato a chiedere il boicottaggio dei negozi ebrei. Proprio ieri, poi, da un sondaggio riportato su un importante quotidiano nazionale, emergeva che il 12 per cento degli italiani si considera antisemita e che nel 44 per cento degli italiani permangono ancora tracce di ostilità. cento condivide gli stereotipi antiebraici che potrebbero definirsi classici nella loro assurdità, come «gli ebrei non sono italiani fino in fondo» e «non ci si può fidare del tutto di loro», «sono vissuti sempre sulle spalle degli altri». Pur trattandosi di un sondaggio, dati come questi devono farci riflettere sulle sacche di intolleranza antiebraica nel nostro Paese e non devono farci abbassare la guardia di fronte al pericolo. Sono sempre più spesso atteggiamenti che trovano i loro padrini politici nell'estremismo di destra e di sinistra. Per questo, le istituzioni del nostro Paese devono reagire a ogni singolo episodio, anche quello che all'apparenza sembrerebbe più marginale. Quando si tratta di antisemitismo, di disprezzo per gli ebrei, dobbiamo proprio in virtù della memoria condivisa, scandalizzarci, indignarci, respingere e reprimere. Sessant'anni dopo quell'indicibile dramma, l'Europa ricorda, ma a volte chiude gli occhi. Non possiamo dimenticare come in altri continenti ancora oggi vengano perpetrati indegni genocidi nel silenzio generale. Sta accadendo ad esempio in Darfur, dove la popolazione viene affamata, stremata, deportata ed uccisa. Oggi siamo chiamati, anche in sede internazionale, a lavorare per un mondo senza genocidi, senza olocausti, che sappia ricordare il dramma della Shoah e quindi non ripeterlo. Signora Presidente, «la memoria umana» - scriveva Primo Levi - «è uno strumento meraviglioso ma fallace». Facciamo in modo che la nostra memoria sulla Shoah non abbia cedimenti e resti sempre viva. Sta a noi custodirla con cura e attenzione, come si fa con la fiamma di una candela per evitare che si spenga.

A nome dell'Italia dei Valori intervengo sul tema che trattiamo avendo ben chiara l'importanza, la gravità e la prospettiva di quello che oggi ricordiamo. È la storia passata, presente e futura dell'umanità che ogni anno ritorna al centro della cultura, della politica e della società intera. Non saranno i nostri interventi, a cominciare dal mio, che cambieranno ciò che è stato, ma abbiamo il dovere di educare le giovani generazioni alla solidarietà e al sano rispetto della persona umana, a qualunque razza appartenga e qualsiasi religione professi. Lo spirito della legge che ha istituito il Giorno della memoria va nella direzione di usare anche questi momenti, questa ricorrenza annuale per riportare alla nostra mente le atrocità di cui l'uomo è stato capace di macchiarsi e per rifiutare i comportamenti che ieri hanno portato persecuzioni e lutti, ma che oggi qualcuno cerca di far rivivere, se non con gli stessi metodi, certamente con gli stessi obiettivi. tutti noi sappiamo che la data odierna è stata scelta perché il 27 gennaio 1945 l'esercito russo entrava ad Auschwitz e mostrava al mondo quanto tutti noi oggi conosciamo. Il primo articolo della legge che istituisce il Giorno della Memoria nel nostro Paese sottolinea come sia un dovere ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), la barbarie delle leggi razziali, la persecuzione dei cittadini di origine ebrea, italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che si sono opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Amare e tutelare il prossimo non è solo un comandamento cristiano, ma è un imperativo laico per preservare l'intera umanità dal desiderio perverso, troppo spesso dietro l'angolo, di assoggettare, distruggere, rubare il futuro ad intere generazioni. Sono stato pervaso da un'intima soddisfazione e da sincera fiducia nel domani apprendendo che in tutta Italia oggi si stanno celebrando tante e tante iniziative ufficiali di ricordo. Ma il ricordo esiste e deve continuare ad esistere anche e soprattutto nei luoghi in cui le coscienze, le idee, i valori universali si formano ed accompagnano l'uomo durante la sua esistenza. Signora Presidente, colleghi, non proseguirò oltre per le intime emozioni che questa ricorrenza mi riporta alla mente: esse appartengono interamente al foro interno di ciascuno di noi, sono una preghiera per il mondo, perché sopravviva all'odio e alla violenza. Voglio solo ribadire l'opportunità di ritenere il Giorno della Memoria un giorno in cui nelle scuole italiane si insegnino ai nostri giovani i principi fondamentali della tolleranza, della cooperazione, della pace. Per questo motivo noi dell'Italia dei Valori chiediamo al Governo

Signora Presidente, il Giorno della Memoria è ormai inciso nella coscienza democratica dei dei popoli e delle Nazioni che, dopo le atrocità naziste, dopo la Seconda guerra mondiale, hanno intrapreso il cammino della libertà e hanno coniugato lo sviluppo economico con il progresso civile.

deportati per motivi politici, ma moltissimi di loro, soprattutto del Nord Italia e nel contesto delle fabbriche, erano semplicemente dei giovani che scioperavano contro il regime perché stanchi della guerra. Tutti questi morti rappresentano una ferita profonda, una ferita che non si rimargina e che, purtroppo, vicende anche recenti riportano in luce nel segno e nel nome di risentimenti e di rancori: i fondamentalismi. È in questo senso che il Giorno della Memoria non si connota come un anniversario rituale, ma sa sempre suscitare forti emozioni e dischiudere la memoria per non dimenticare. è il peggiore nemico di chi voglia cercare riscatto e soprattutto evitare per il futuro quelle turpi pagine che sono la macchia più buia del XX secolo. secolo. Ma non basta ricordare, non è sufficiente leggere i libri di storia: occorre allenarsi al rispetto dell'uomo in tutte le sue espressioni, in una dimensione di reciprocità, di mutuo riconoscimento delle singole peculiarità. È con questo spirito che non celebriamo la Shoah, ma la eleggiamo a silenziosa lezione di questa giornata carica di dolore, ma ricca di insegnamenti. Signora Presidente, onorevoli colleghi, sarà l'improvvisa crisi finanziaria ed economica che ha coinvolto tre quarti del pianeta, l'eco delle bombe e dei razzi su Gaza e Israele, la coinvolgente lezione di Obama, il diffondersi di violenze contro le persone più indifese (a cominciare dalle donne), il concitato momento in cui versa la questione degli immigrati: sarà questo o altro, sta di fatto che siamo arrivati al Giorno della Memoria un po' svuotati dell'empito da cui nacque. Abbiamo a tal punto banalizzato la vita e la morte che ciò può accadere anche per la storia, la quale parla sempre più da lontano. Eppure, nella vita dell'umanità c'è un passato che non è mai passato del tutto e non possiamo accettare le ottuse o subdole pretese di cancellarlo. Ecco perché il nostro Parlamento, su iniziativa del senatore Furio Colombo, votò all'unanimità l'istituzione del Giorno che si sta celebrando. Siamo come ingrigiti nel troppo tempo concesso alla dimenticanza, all'ambiguità, all'arrendevolezza, persino alla menzogna. Bisognerebbe costringere la storia a restare sotto i nostri occhi, se del caso criticandola, sbugiardandola, additandola, non per far durare il rancore - dal momento che ci è impossibile zittire una voce anche cristiana, fondata sulla pietà - ma perché non muoia la certezza della colpa e la lezione della sofferenza. Sebbene milioni di uomini abbiano avuto la vita rubata, sfigurata, incenerita, un grande salto generazionale ha disteso una sorta di oblio sull'onta del secolo. Non è più tempo di memoria, si sente dire. Essa attarda il presente e allontana il futuro. A tale processo, che ha qualcosa di indicibile, ha messo mano chi, avendo dell'esistenza e della storia un sentimento quotidiano e indistinto, vorrebbe liberarsi da ogni responsabilità precedente. Non mi richiamo all'abusata, declamatoria saggezza secondo la quale chi non sa giudicare il proprio passato è destinato a riviverlo: dico, semplicemente, che una così grande tragedia esige di non essere dimenticata in un tempo che, secondo l'analisi di uno storico apocalittico, si avvia a diventare «una continua rincorsa tra l'informazione e la catastrofe». Ma «un uomo è un uomo per il suo avvenire», ha scritto Borges, e non potremmo affrontarlo senza la nozione di ciò che siamo stati e di come abbiamo agito. Chissà se, nel togliersi la vita, Primo Levi è stato assalito dal frastuono o dal silenzio della sua vita. «Un uomo che è stato torturato rimane torturato», aveva detto.

«Senza il ricordo non siamo nulla, non resta che aspettare l'amnesia finale, che cancella una vita intera». Signora Presidente, sono trascorsi sessantaquattro anni, come ha ricordato poco fa presidente Schifani, da quando un'avanguardia dell'esercito americano entrava nel campo di Auschwitz e il filosofo Theodor Adorno disse che non sarebbe stato più possibile scrivere una poesia. Forse non era un allarme soltanto morale: egli si pronunciava anche contro l'«estetizzazione» della sofferenza, giudicandola un modo di trasferire i contenuti dentro la cornice dell'enfasi e del dolorismo, anziché lasciarli a un giudizio nudo, fondato sulla storia. Questa tesi mi è parsa chiara ascoltando, nella trasmissione «I giorni e la storia», un'anziana signora che aveva perduto a Dachau dodici tra familiari e congiunti ed era sfuggita, non si sa come, alla camera a gas: essa dichiarava di voler vivere a lungo perché, disse, morto chi vide, nessun altro, neppure il più reputato degli storici, o degli scrittori, o dei poeti, potrà rendere credibile quel crimine. Un giorno, temeva la donna, tutto rimarrà affidato alle volenterose, ma incredibili rievocazioni ideologiche, alle rappresentazioni drammaturgiche, se non addirittura agli ingenui racconti dei cantastorie. Un grande salto generazionale, inedito nella sua irrevocabilità, sta infatti cancellando vita e morte di chi conobbe l'onta del secolo. Oggi il mondo ha una memoria che comincia al di qua di quell'immane peccato. Eppure abbiamo ancora tremendi motivi per dire che la memoria non è una sbiadita coscienza che ha già concluso il suo cammino, ma ciò che tiene in vita proprio quella coscienza; perché il ricordare, nel senso che qui oggi intendiamo, è un dovere etico, e farne passare il significato di generazione in generazione è una pedagogia paterna, nutrita da un amore fatto di carne e spirito, che scorre lungo le vene di una filiale continuità, prima ancora che sulle pagine dettate dalla storia. Ho incontrato, nel mio lavoro, diversi giovani che esprimevano una volontà dissacratoria rozzamente declamata, ma che non poteva non essere l'avvisaglia di qualcos'altro, un'imprecisa inquietudine che si placava solo volgendola in rancore, intolleranza, violenza; e che cercava un tratto sciagurato d'identità nei simboli presi dai repertori non solo della stupidità, dando la sensazione di voler sputar fuori qualcosa di oscuro e di minaccioso. In realtà, tutto insorgeva da un vuoto di conoscenza pari soltanto all'incapacità di capire; dove però l'imbecillità si appassionava e c'era sempre più d'uno che fingeva di credere in qualche, seppur truce, oltre che malinteso, ideale. Da allora abbiamo continuato a leggere sui muri di città e paesi, stadi e scuole, chiese e cimiteri la loro prosa sciagurata e nondimeno ascoltato la discolpa della loro età, se non addirittura della loro innocenza, da un altro sventurato versante: quello di un insorgente negazionismo. Persino un vescovo lefebvriano ha avuto, come oggi titola a tutta pagina «l'Unità», «un vuoto di memoria». Con queste premesse non dovremmo informare i giovani riandando a ciò cui ci richiama la memoria? La loro coscienza non dovrà essere avvertita di fronte al perdurare, addirittura all'aggravarsi, di ciò che dovrebbe invece ammonirli? Certo, non dovrà venir meno la costante e laboriosa disposizione della democrazia a trarre da queste temperie motivi di riflessione rigorosa e ferma, anziché rabbie emotive o sterili sdegni; e alla famiglia, alla scuola, ai *mass media*, al Parlamento, alla Chiesa spetterà, piuttosto, di fare ciascuno la propria parte, per essere instancabili eredi e continuatori del ricordo in quanto strumento di una rinnovata consapevolezza. Ciò per vivere una rigenerazione civile e spirituale, secondo il principio in base al quale la ragione non può stancarsi di ragionare. Proiettare la memoria nel futuro non dev'essere un perdurante, sfiduciato, pessimistico sentimento di insicurezza, ma un segno di civismo, di moralità, di avvedutezza. Chiudere un libro, insomma, ma tenendo aperta l'ultima pagina, quella del bilancio e della previdenza, che stanno - come sempre nella vita - tra passato e futuro. In ciò sorretti dalle parole di Agostino d'Ippona, il quale dice: «Da due pericoli dovremo ugualmente guardarci, dalla disperazione senza scampo e dalla speranza senza fondamento». Elias Canetti darà un volto laico, per dir così, a questa speranza. Egli dice: «Certe speranze, quelle pure, quelle che nutriamo non per noi stessi, quelle il cui adempimento non deve tornare a nostro vantaggio, le speranze che teniamo pronte per tutti gli altri, che procedono dalla bontà innata della natura umana, poiché anche la bontà è innata, queste speranze di un giallo solare bisogna nutrirle e difenderle quand'anche non dovesse mai giungere l'istante in cui si compiano: perché nessun inganno è altrettanto sacro, e da nessun altro dipende a tal punto la nostra possibilità di non finire completamente sconfitti». Uno storico ha immaginato che questo tempo stia inaugurando un fenomeno fino a ieri impensabile: la cronaca, per effetto della velocità impressa dalla comunicazione, è ormai contigua alla nostra storia. E la memoria comincerebbe solo dall'altro ieri. Non credo che ciò accadrà presto, ma occorre fin d'ora persuaderci che il pericolo è sempre meno il pericolo e sempre più la mancata percezione del pericolo. Una saggezza da poco, direte: la questione, è vero, esigerebbe molto di più. Ma «tutto, della storia» - ha detto Toynbee «a veder bene comincia ogni giorno dal poco». «Perciò» - ha aggiunto - «ogni uomo, anche il più semplice e debole, è tutta l'umanità». Uno di quei giorni è oggi, ed è di tutti.

ricordando lo sterminio perpetrato dai nazisti e rivelato al mondo sessantaquattro anni fa, non si può che ripetere il "mai più" tante volte pronunciato, tante volte udito in queste giornate della memoria. Chi mai potrebbe, almeno fra coloro che hanno una scintilla di ragionevolezza e di umanità, non rifiutare in modo integrale l'abisso e la malvagità di Auschwitz, i 6 milioni di ebrei sterminati, milioni di uomini, di donne, di bambini e bambine cui non fu tolta soltanto la vita? Gli assassini, infatti, tentarono di privarli di qualunque cosa li rendesse umani: tolsero loro i nomi, sostituiti da un numero; tolsero loro le famiglie, smembrate secondo logiche organizzative; tolsero ogni effetto personale; tolsero persino i corpi, da vivi trasformati in macchine al servizio dello sforzo bellico, e da morti smaltiti come fossero merce o addirittura rifiuti. I sopravvissuti raccontano che quando ad Auschwitz furono messi in funzione i forni crematori il comandante diede l'ordine di riesumare le migliaia di cadaveri che in precedenza erano stati seppelliti in massa, allo scopo di bruciare anche questi. un'altra scelleratezza veniva imposta ai prigionieri che facevano questo terribile lavoro: a loro, che in quei resti spesso riconoscevano le sembianze di un familiare o di un amico, era proibito chiamarli corpi o cadaveri, quali erano; dovevano chiamarli figure o pupazzi. In quest'orrendo episodio sta forse proprio l'opposto di ciò che questa giornata si propone. Ciò che gli assassini tentavano di nascondere o di far dimenticare, noi dobbiamo svelarlo e ricordarlo; ciò che volevano negare e chiamare con un nome falso, dobbiamo portarlo ancora alla luce della verità. Chi oggi non condivide la memoria della Shoah come monito a che mai più si ripeta una cosa simile usa in fondo le stesse tecniche di quel comandante scellerato: comandante scellerato: far scomparire la verità, o negandola, o chiamando le cose con un nome falso, perché la verità sarebbe stata impossibile da accettare persino per i più fanatici dei nazisti, ai quali, pure, era stato insegnato a odiare e disprezzare nel massimo grado tutti gli ebrei. Così succede anche oggi. Gli odiatori degli ebrei tendono a usare due mostruosità insieme che si contraddicono a vicenda: per un verso negano la Shoah, uccidendo ancora una volta le sue vittime; per un altro ne auspicano la ripetizione e ne osannano gli autori, mascherandola con motivi più adatti ai tempi, con nuovi nomi. Non propugnano più l'odio per gli ebrei in quanto deicidi, ma in quanto ricchi e potenti capitalisti e finanzieri; non propongono più di far piazza pulita del ghetto della città, ma di distruggere lo Stato di Israele; non parlano più, almeno in Occidente, dei Protocolli dei Savi di Sion o di sacrifici umani perpetrati durante le cerimonie ebraiche,

non parlano più di eliminare la razza ebraica perché non contamini una qualche presunta razza superiore, ma auspicano che Israele sparisca e cessi finalmente di minacciare la pace, come intendono in parecchi. A tutto questo e a molto altro oggi dobbiamo dire "mai più" ricordando quello che accadde. Lo sterminio degli ebrei non fu un'idea che venne a Hitler una volta preso il potere o una volta iniziata la Seconda guerra mondiale. In un'intervista del 1921, quando era soltanto l'oscuro *leader* di un partitucolo di reduci frustrati, di disperati pieni di paura e di risentimenti, ad un giornalista che gli chiedeva cosa avrebbe fatto se avesse vinto le elezioni in Baviera, dove agiva in quel periodo, rispose che avrebbe messo una o due forche nella piazza centrale di Monaco e avrebbe impiccato tutti gli ebrei. Non lo presero sul serio, a cominciare dal giornalista che lo intervistava, ma sbagliarono. Anche oggi c'è chi fa proclami del genere, Ahmadinejad e Hamas per esempio, ma si preferisce ritenere che siano, tutto sommato, intemperanze verbali, che siano paroline scappate in un momento di entusiasmo. È accaduto anche con altre vittime: Pol Pot prometteva di eliminare la classe borghese dalla Cambogia e tanti, in piazza e in certi congressi, inneggiavano a lui, che poi fece esattamente ciò aveva promesso, uccidendo un terzo dei suoi connazionali. Allora, mai più non prendere sul serio chi lucidamente e ripetutamente promette morte e distruzione. Poi quell'oscuro attivista politico divenne il capo indiscusso della Germania e quando avanzò pretese irragionevoli verso i vicini, in particolare i cechi, i grandi *leader* europei corsero a convincere il povero presidente Benes ad accettare le intimazioni che gli venivano da Hitler, in nome della pace, della tranquillità e del quieto vivere. Un anno di pace che Hitler usò per impadronirsi di nuovi territori, armarsi, preparare la guerra mondiale e lo sterminio degli ebrei. Allora, mai più piegarsi alla prepotenza e alla violenza con il risultato di incoraggiare l'una e l'altra. Gli ebrei nell'Europa degli anni '30 - ma anche oggi - venivano accusati perché facevano esattamente ciò che facevano tutti: cercare di migliorare la propria situazione economica praticando le attività che era loro possibile. Poiché per secoli era stato loro proibito di coltivare la terra, erano particolarmente attivi in quello che noi oggi chiamiamo terziario, attività che proprio in quel periodo si rivelò la più redditizia. Di qui l'invidia, il risentimento, l'odio, poi i *pogrom* e la Shoah. Oggi Israele fa ciò che fa qualunque Stato: si difende da chi lo attacca. Fin dal giorno in cui fu fondato, è stato oggetto di ripetuti attacchi.

reagire. Allora, mai più applicare agli ebrei o al loro Stato un metro diverso da quello che si applica a tutti. oggi rispetto ad allora molto è cambiato: sono cambiate le divise di chi diffonde l'odio, sono cambiati gli slogan, sono cambiate le menzogne, sono cambiate le ragioni per cui si attaccano gli ebrei. Negli anni '30 in Germania lo si faceva per una perversa e degenerata forma di orgoglio per la propria Nazione, nell'Inghilterra di oggi si toglie la Shoah dai libri di scuola per un malinteso e perverso senso di tolleranza e di rispetto verso coloro che non hanno piacere di sentire questi argomenti. Allora, il nostro "mai più" oggi, perché sia davvero vivo e operante, deve essere un no contro ciò che era vero allora ed è vero oggi, cioè che la malvagità e l'odio, che sempre sono intrecciati alla menzogna, alla malvagità e all'odio di pochi, uniti all'indifferenza dei milioni di persone, degenerare in un abisso. Dire "mai più" significa combattere e contrastare l'odio, ma anche combattere e contrastare l'indifferenza.

Do la parola al presidente della 5a Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria del decreto-legge al nostro esame. *(PdL)*. Signora Presidente, la Commissione bilancio ha preso in esame i profili di copertura finanziaria connessi alla questione di fiducia posta dal Governo. A seguito delle risposte articolate che sono state date sui vari punti che la Commissione aveva preso preso in esame, considerato anche che il Governo ha fornito una tabella puntuale - in termini tecnici un allegato 7 molto preciso - che evidenzia il non peggioramento dei saldi, la Commissione ha preso atto di tutto questo con evidente

*(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo a votare l'ennesima fiducia ad un Governo che gode di una maggioranza tra le più larghe dell'intera storia repubblicana: di nuovo il Senato è espropriato della sua prerogativa costituzionale di dibattere liberamente i provvedimenti dell'Esecutivo; di nuovo si umilia il Parlamento, impedendo ai parlamentari di entrare nel merito dei provvedimenti e di proporre modifiche migliorative. Speravamo, dopo l'esperienza positiva del disegno di legge sul federalismo fiscale, che si proseguisse sulla strada del confronto, l'unica che può portare benefici al Paese, soprattutto in momento drammatico per la nostra economia nazionale, un momento che obbligherebbe a scelte forti e condivise. E invece no, avete preferito, ancora una volta, la contrapposizione. Nel merito, il provvedimento in esame è del tutto inadeguato a rispondere alla gravità della crisi economica che si acuisce giorno dopo giorno. È di oggi l'ultimo allarme, quello dell'amministratore delegato di FIAT Marchionne, sul pericolo occupazione per 60.000 lavoratori del settore auto. Non si contano le aziende in crisi, mentre esplode il ricorso alla cassa integrazione. In questo scenario, il Governo non è in grado di mobilitare risorse adeguate. Il Paese paga a caro prezzo le scelte sciagurate, da cicala imprevidente, fatte all'inizio della legislatura: l'esenzione totale dell'ICI per i ceti abbienti

del loro risparmio? Anche queste sono diventate, evidentemente, carta straccia. In totale, parliamo di 5-6 miliardi, che oggi sarebbero molto utili per dare sollievo a coloro che perdono il lavoro, i precari *in primis*, al crescente numero di cittadini bisognosi, e per sostenere le imprese nello sforzo di rinnovamento necessario per il proprio rilancio produttivo. In particolare, è esiguo l'impegno nel campo delle infrastrutture. Tutti i Governi del mondo hanno deciso di investire risorse importanti nelle infrastrutture materiali ed immateriali, considerate giustamente la parte decisiva delle politiche anticicliche, da Obama a Sarkozy, dalla Merkel a Brown. Da noi no; da noi non si riesce neppure a trovare le risorse per avviare le opere già approvate dal CIPE. Nonostante i tanti ordini del giorno, anche unitari, il Governo non si muove. La borsa del ministro Tremonti, vero *deus ex machina* dell'Esecutivo, rimane ermeticamente chiusa. E allora non partono le opere previste per Expo Milano 2015, non parte l'Alta velocità sulla Milano-Verona e sulla Milano-Genova, né partono tante altre opere. In questo modo, temiamo che l'Italia rischi di uscire dalla crisi molto peggio di come vi entra, senza cioè aver realizzato quelle opere strategiche che tutti giudicano essenziali come volano per l'oggi e come *condicio sine qua non* del rilancio competitivo del Paese. Così non va. L'articolo 25 dà una boccata d'ossigeno alle Ferrovie dello Stato, con 960 milioni di euro, ma è giusto ricordare che la finanziaria aveva ridotto di un terzo le risorse assegnate dalla precedente finanziaria del Governo Prodi alle nostre ferrovie dello Stato. Si tratta perciò di un necessario provvedimento correttivo, ma limitato, che non riuscirà ad invertire la tendenza al declino del nostro trasporto ferroviario,

Il comma 2 destina 480 milioni al trasporto regionale. Anche in questo caso, rispetto ai bollettini di guerra provenienti dalle varie regioni sulla situazione dei treni dei pendolari, riteniamo che questo provvedimento non riuscirà a sanare né i guai antichi né quelli nuovi. Si tratta di risorse del tutto insufficienti. Noi crediamo, invece, che serva un piano straordinario, che consenta finalmente ai pendolari di poter disporre di un servizio all'altezza di un Paese civile. La Camera ha modificato col cosiddetto emendamento salva Malpensa l'articolo 19. Si tratta di un primo passo nella giusta direzione: quello della liberalizzazione dei diritti di volo per le rotte intercontinentali, ma non è la panacea di tutti i mali che affliggono Malpensa. Ci vorranno anni di negoziati internazionali per avere i primi risultati. Nel frattempo nulla si fa per dare una risposta al punto critico numero uno dello scalo varesino, l'accessibilità. Le opere che consentirebbero di connettere l'aeroporto all'Alta velocità Torino-Milano e con la stazione Centrale di Milano non vengono finanziate, così come non viene risolta la questione cargo. cento delle merci da e per l'Italia passavano da Malpensa e ora questo servizio è cessato. La Camera di commercio di Monza ieri ha illustrato uno studio che prevede un danno di 2 miliardi e mezzo per le imprese lombarde proprio per l'impossibilità di far viaggiare le merci, che oggi vengono caricate sui camion e portate a Parigi o ad Amsterdam per essere poi spedite in aereo in America o in Asia. Questa è la nostra *green economy*: mettere le merci sui camion. Gli altri fanno investimenti importanti, noi, invece, azzoppiamo un aeroporto come quello di Malpensa e torniamo al vecchio metodo appunto dei camion. Complimenti: un vero aiuto alle imprese in difficoltà! Da ultimo mi consenta, Presidente, un breve commento sull'articolo 31, che aumenta l'IVA sulle tv satellitari. Che sia un provvedimento anti SKY è indubitabile; non si può accampare il pretesto dell'armonizzazione fiscale richiesta dall'Europa, non c'era nessuna infrazione formale e quindi nessuna urgenza. La realtà è più semplice. In una fase di forte competizione tra le piattaforme televisive e tra i *broadcaster* si penalizza uno dei competitori e una piattaforma, quella satellitare, a tutto vantaggio della *pay tv* sul digitale terrestre che - guarda caso - è della azienda del Presidente del Consiglio. Ancora una volta siamo in pieno conflitto d'interesse. Per tutte queste ragioni e per il netto giudizio politico negativo sul provvedimento in discussione, il Partito Democratico voterà no alla fiducia chiesta dal Governo.

il senatore Paravia ci ha detto che, se il Governo avesse posto la fiducia, oggi avremmo ascoltato in questa Aula le solite grida sulla mortificazione del Parlamento, grida magari piene di ipocrisia e di enfasi. Ora che la fiducia è stata effettivamente posta, io invece non mi rassegno, non mi voglio rassegnare a considerare come semplice esercizio di retorica e di ipocrisia il fatto di sottolineare, ancora una volta, la degenerazione del rapporto tra Governo e Parlamento, che in modo sistematico sta caratterizzando questi mesi di legislatura; di denunciare, ancora una volta, che per il numero dei decreti-legge, per la rilevanza e la complessità delle materie che sono state affidate agli strumenti della decretazione d'urgenza e del voto di fiducia, questo Parlamento è stato ridotto ad una funzione di ratifica delle decisioni assunte altrove. rimarcare che l'atteggiamento serio e responsabile del Gruppo del Partito Democratico, sia alla Camera che al Senato - dove non è stata messa in atto alcuna azione ostruzionistica, dove il numero degli emendamenti presentati avrebbe permesso comunque l'approvazione del provvedimento entro i termini previsti, dove vi è stata la nostra disponibilità al confronto sulle misure da adottare per affrontare l'emergenza - ha fatto emergere affrontare l'emergenza - ha fatto emergere in modo chiaro che le difficoltà stanno tutte al vostro interno e che non siete riusciti a tenere insieme le vostre non piccole contraddizioni. E non è in gioco soltanto la dignità dell'opposizione, anche perché, oggi, c'è un motivo in più per esprimere tutto il disagio politico e istituzionale per questa porta sbarrata a qualsiasi tipo di confronto di merito. Ed è il fatto che l'oggetto di questo decreto-legge è la crisi, quella crisi che sta interrogando e sfidando i Governi a trovare modi, misure e strumenti per arginarla, per invertire la tendenza di un ciclo recessivo che non ha precedenti nella storia del mondo moderno, quella crisi che nel mondo sta mettendo in discussione i fondamentali dell'economia. «Ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», così recita il titolo del provvedimento: se solo ci fermiamo per un attimo al significato di queste parole, è sconcertante il divario tra l'obiettivo e il contenuto reale. Così come è sconcertante l'abisso tra propaganda e realtà. Il Governo ha sbandierato solo pochi mesi fa che avrebbe messo 80 miliardi in campo per superare la crisi, ed è finita con questi miseri 5 miliardi. Ha sbandierato che sarebbe intervenuto a favore delle famiglie, soprattutto quelle con figli perché più in difficoltà, ed è finita con un *bonus una tantum,* che per la gran parte è destinato a *single* e coppie senza figli, introducendo di fatto un coefficiente familiare al contrario e con una clamorosa svista - chiamamola così - sui portatori di *handicap*. ha sbandierato la difesa dei più deboli, vestendo i panni di Robin Hood, ed è finita con un raggiro clamoroso e mortificante nei confronti dei più bisognosi; non perché a noi non vadano bene i 40 euro al mese, ci mancherebbe! Il problema è che li prendano, il problema è che devono sottostare a procedure burocratiche complicatissime ed oltretutto costose per il Paese.

Chi sarebbe allora *radical chic*? Ieri tutti gli interventi dei colleghi del mio Gruppo, concentrandosi ognuno su temi diversi, hanno argomentato con ampiezza le ragioni del nostro dissenso su questo provvedimento, che stanno soprattutto nel vuoto di risposta, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, delle misure predisposte dal Governo. Il Governo non è stato sin qui all'altezza della drammaticità della situazione che abbiamo di fronte. di stipendi, salari e pensioni, al tessuto produttivo, agli enti locali, a chi oggi ha perso o sta perdendo il posto di lavoro, non ci è permesso di dire: vedremo, abbiate fiducia, siate ottimisti, mal che vada si ritorna alla situazione del 2006. Cosa diciamo invece a loro adesso, ora, quando su tutti i giornali leggiamo dei 60.000 operai a rischio nel comparto auto, quando sui giornali locali continua il bollettino di guerra delle difficoltà delle aziende nei nostri territori? Se il 2009 vedrà il nostro Paese dover far fronte ad una cifra variabile tra i 500.000 e il milione di disoccupati, cioè donne e uomini, giovani, famiglie che improvvisamente perdono il lavoro, di fronte ad un impatto improvviso così violento, tale da mettere in crisi il nostro sistema di ammortizzatori sociali e soprattutto il nostro sistema di coesione sociale, chi oggi prova a dividere i lavoratori e le loro organizzazioni commette un errore enorme. Questo Paese si salva e si può rimettere in moto se vi è una politica che unisce, se vi è una classe dirigente che si assume la la responsabilità di costruire una visione comune, un progetto, se si fanno le riforme necessarie a far funzionare meglio le cose, anziché giocare la partita, tutta politica, della divisione tra i sindacati. Per noi l'unità delle forze del mondo del lavoro è un bene in sé, tanto più per fronteggiare un momento così difficile sul piano economico e sociale. Abbiamo detto più volte, e l'abbiamo dimostrato con l'assoluta responsabilità del nostro atteggiamento e del merito delle nostre proposte, che il Partito Democratico era pronto a dare un contributo su questi temi. Ma servirebbe un Governo disposto ad un confronto diverso con l'opposizione, un Governo più attento alla funzione del Parlamento, meno attento ai sondaggi, ai titoli dei giornali e più attento invece alle persone in carne ed ossa, ai loro problemi ed alle loro necessità. da tutta questa vicenda emerge una verità indiscutibile: avete i numeri per essere maggioranza, ma non la compattezza per votare i vostri provvedimenti senza ricorrere al voto di fiducia. In campagna elettorale si può dire tutto e il suo contrario; dopo, no: bisogna governare, trovare le soluzioni e fare i fatti, non solo propaganda. E voi, certo bravi nella propaganda, alla prova dei fatti state dimostrando tutta l'inadeguatezza e l'irrilevanza delle vostre scelte.

con la fiducia messa dal Governo - sia alla Camera, sia al Senato - su questo provvedimento è stata sottratta al Parlamento per l'ennesima volta la possibilità di discutere e prendere decisioni efficaci su questioni di primaria importanza, quale quella della crisi economica che sta attraversando il nostro Paese. Addirittura, in Commissione lavoro, in maniera assolutamente irrituale, abbiamo espresso il parere su un provvedimento, il milleproroghe, che contiene al suo interno norme recanti interventi su materia identica a quella disciplinata dal provvedimento sul quale oggi siamo chiamati a votare la fiducia e di cui non abbiamo avuto la possibilità di discutere. Questo per sottolineare quanto questa maggioranza tenga in considerazione il lavoro parlamentare e il parere delle Commissioni. Non voglio comunque rinunciare a far rimanere agli atti dei lavori di quest'Aula almeno quello che il Gruppo dell'Italia dei Valori in tema di lavoro avrebbe voluto modificare, se ci fosse stata la possibilità di svolgere un vero confronto, per rendere questo provvedimento *spot* un po' più credibile, visto che così com'è è assolutamente insufficiente a fronteggiare una crisi di portata mondiale come quella in atto. In materia di lavoro, il problema cruciale cui far fronte in questo momento di grave crisi è la caduta del potere d'acquisto di salari e pensioni ed il conseguente drastico peggioramento del tenore di vita dei percettori di tali redditi, situazione è aggravata dalla presenza di contratti di lavoro precario. Per questa ragione, avevamo presentato un emendamento all'articolo 1 del decreto, volto a trasformare il *bonus* previsto in un aumento degli assegni al nucleo familiare, rendendo permanente la misura, in modo da incentivare realmente i consumi e riequilibrare il carico fiscale a carico delle famiglie. Sempre all'articolo 1, avevamo introdotto la costituzione di un fondo per il sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, per gli anni 2009 e 2010, le cui risorse sarebbero state destinate alla riduzione permanente del prelievo fiscale sui redditi da lavoro dipendente e da pensioni inferiori a 35.000 euro annui, attraverso l'aumento delle detrazioni. Avevamo presentato un emendamento all'articolo 2, comma 5, che prevedeva un'autorizzazione di spesa finalizzata ad aumentare l'importo degli assegni familiari previsto, in modo da avere una copertura reale e non proveniente dall'eventuale risparmio dei fondi per il sostegno ai mutuatari in difficoltà. Ancora, l'emendamento all'articolo 4 proponeva che i contributi previdenziali per il lavoro dei volontari del servizio civile rimanessero a carico del Fondo nazionale del servizio civile. Ma, soprattutto, all'articolo 19 avevamo presentato emendamenti volti a dare un sostegno reale ai lavoratori, perché quanto previsto dallo stesso articolo sugli ammortizzatori sociali rappresenta solo un intervento tampone, che nulla ha a che vedere con le reali esigenze del nostro Paese. I lavoratori, costretti a fronteggiare condizioni di vita sempre più difficili, necessitano di una diversa politica salariale e un deciso rilancio del *welfare* pubblico. Per quest'ultimo, però, assistiamo per l'ennesima volta all'immancabile evocazione dell'attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, aspettando la quale si provvede con il consueto provvedimento tampone, ovvero con l'abusata misura della concessione degli ammortizzatori in deroga. Per questo proponevamo, sul modello tedesco, il pagamento da parte dello Stato delle ore non lavorate per i dipendenti delle aziende in crisi che riducano gli orari di lavoro senza licenziare, mettere in cassa integrazione o in mobilità i propri dipendenti, incrementando le risorse del del Fondo per l'occupazione di 700 milioni di euro annui. Sempre in questo articolo, viene introdotta una prima forma embrionale di indennità di disoccupazione per i Co.co.co, che proponevamo di estendere anche ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e così via. A causa della crisi, il quadro lavorativo in Italia andrà sempre più peggiorando. I lavoratori precari in Italia sono circa 3 milioni e a molti e a molti di questi nel 2009 non verrà rinnovato il contratto. La vera emergenza, nei mesi a venire, sarà questa e la sfida per il Governo e per tutti noi sarà dare risposta a questi lavoratori e alle loro famiglie, che presto saranno travolti dalla crisi. Come fate, mi chiedo, a dare così pochi soldi ai lavoratori italiani, quando darete 5 miliardi di dollari alla Libia, con il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia tra il nostro Paese e la Libia?

in cui si registra una profonda sfiducia da parte dei cittadini verso le istituzioni. Proprio in questo momento, il Governo avrebbe dovuto dare una risposta rassicurante

In questo breve intervento cercherò di sviluppare un argomento specifico, dal momento che molti colleghi, prima di me, hanno analizzato nel dettaglio il provvedimento.

nel testo è non solo dimenticata, ma soprattutto offesa. L'iniziale mancanza di una politica strutturale familiare si è tramutata nell'urgenza di un decreto che, pur essendo necessario,

dagli organi di informazione, non saranno le famiglie a beneficiare di questo intervento, oltretutto *una tantum*, ma per l'82 per cento se ne avvantaggeranno *single* e coppie senza figli. Se correttamente - e ce lo dicono tutti gli studiosi - si volevano privilegiare le famiglie con figli, dal momento che i dati dimostrano che sono le più incapienti, allora serviva almeno un correttivo: prescindendo dalla relazione e dalla stabilità del legame affettivo, la presenza di uno o più figli doveva consentire la percezione dello stesso *bonus*. Questo decreto pasticciato e confuso

La nostra legislazione ha riconosciuto la parità di diritti tra figli di una coppia di fatto e figli nati in costanza di matrimonio. Fortunatamente, a tale riguardo la nostra legislazione ha fatto giustizia. in esame, però, si attua una discriminazione *a contrario*, in quanto i primi vedranno i genitori percepire due *bonus*, mentre i secondi rischiano di essere addirittura esclusi, che il reddito dei loro genitori sarà cumulato; eppure vivono con lo stesso identico reddito. Questo per dimostrare l'ingiustizia, l'assurdità di quanto Il messaggio che si evince da questo provvedimento è un terribile segnale che mina l'assunzione di responsabilità nelle relazioni affettive. I giovani capiscono e lo capiscono molto bene - che è più vantaggioso economicamente non sposarsi. Era sufficiente un piccolo correttivo per riparare a questa ingiustizia, ma il Governo ha ritenuto opportuno non intervenire: non è intervenuto alla Camera e non interviene qui al Senato. una vera ingiustizia sociale questa che viene operata; per operare invece una giustizia sociale si sarebbe dovuto rivedere la parametrazione, perché quest'ultima fotografa la realtà. Non dobbiamo illudere le famiglie. Su questo credo che anche alcuni colleghi della maggioranza dovrebbero essere d'accordo. Anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel suo tradizionale

Concludo affermando che la centralità della famiglia per questo Governo serve solo per gli *spot* elettorali, perché quando si tratta di fare politiche concrete il centrodestra è terribilmente *single*.

l'epilogo a cui sta giungendo questo provvedimento è quanto di più sbagliato e dannoso si potesse immaginare in questa fase difficile per il Paese e per la situazione di difficoltà in cui vengono a trovarsi un numero sempre maggiore di nostri concittadini e le loro famiglie. Avere chiesto la fiducia su un provvedimento che riguarda l'approvazione di misure relative al futuro del lavoro, dell'occupazione, della tenuta del nostro sistema produttivo e degli interventi a sostegno delle famiglie è un gesto di divisione del Paese ed il perseguimento di un atteggiamento di contrapposizione, che è l'esatto contrario di ciò di cui avremmo bisogno per affrontare una crisi difficile e di non breve durata. Voi continuate a dividere invece di unire gli sforzi per affrontare in maniera solidale le sfide e le incognite che stanno di fronte a tutti. Non è il contributo costruttivo dell'opposizione ciò che state cercando nel Parlamento e nella società. D'altronde, il Presidente del Consiglio, che invoca la leggerezza quando affronta con battute da caserma il sentimento di orrore e di disprezzo che provano le donne verso la recrudescenza della violenza nei loro confronti, ha paura di ammalarsi di itterizia se ascolta e tiene conto delle proposte concrete che provengono dal nostro partito e dalle altre forze di opposizione. Tempi difficili per riportare alla ragione e alla responsabilità chi più di altri dovrebbe invece cercare di raccogliere le proposte, i suggerimenti e le forze migliori per far fronte ad una crisi che sta già producendo effetti devastanti in vaste aree del Paese e soprattutto tra i più deboli ed i meno tutelati: gli anziani, gli indigenti, i giovani e i precari, le donne che vedono venir meno i servizi sociali e il lavoro. Voi continuate la vostra opera di divisione: i forti contro i deboli, il Nord contro il Sud, gli italiani contro gli immigrati regolari e non, perché dovete trovare un nemico, o più di uno, a cui addebitare ciò che si sta delineando ancora una volta e cioè la vostra incapacità a governare questo Paese, al di là dei consensi elettorali ottenuti sull'onda di promesse che non riuscite a mantenere, e di paure alle quali non siete in grado di dare risposte rassicuranti e durature. Anche la divisione sindacale che avete perseguito ed assecondato è figlia dell'incapacità a svolgere un ruolo di governo e di composizione dei conflitti, anzi la vostra è una cultura che vive e si alimenta dalla sistematica emarginazione di tutti coloro che considerate avversari della vostra infallibile ricetta di presunta modernità. Questi sono errori che pagheremo cari, non solo chi vi ha dato il consenso, ma l'intero Paese che è costantemente sospinto, irrazionalmente, verso una deriva populistica e massimalista che non consente di adottare con coerenza tutti quei provvedimenti necessari per affrontare con decisione una crisi che non è solo di ordine economico, ma è una crisi di valori, di solidarietà, di appartenenza ad un destino comune. In quest'Aula qualche giorno fa è passato un provvedimento, quello sul federalismo fiscale, che nel metodo - e per certi aspetti anche nel merito - ci aveva fatto sperare in un atteggiamento diverso e di maggiore attenzione alle proposte che provenivano da parte di un'opposizione responsabile, quale noi siamo, che è impegnata a dare risposte positive ai bisogni dell'intero Paese. Il numero molto limitato dei nostri emendamenti lo dimostra, diversamente dal trattamento che voi avete riservato al precedente Governo guidato da Romano Prodi. Non avevamo però tenuto conto che il vostro Governo e la vostra maggioranza affrontano le proprie contraddizioni sistematicamente con le doppie verità, pur di rimanere assieme, uniti dal collante di un potere fine a se stesso. Prima di me i miei colleghi ne hanno ripercorse molte. Per quanto mi riguarda mi soffermerò, a questo punto, solo su due temi che gettano un'ombra significativa sulla coerenza tra ciò che è stato approvato la settimana scorsa in tema di federalismo e ciò che state per affrontare con questo decreto. Mi riferisco in primo luogo alle politiche di sostegno e sviluppo del trasporto pubblico locale. nonostante il trasporto pubblico locale si sia convenuto essere uno dei servizi essenziali da erogare ai cittadini, e in particolare ai pendolari, agli studenti, alle persone anziane e a tutti coloro che non dispongono o non possono utilizzare un mezzo proprio, nel decreto-legge viene indicato un finanziamento di soli 30 milioni di euro, Le imprese ferroviarie regionali sono contestualmente del tutto dimenticate, escludendole sia dal finanziamento erogato a Ferrovie dello Stato-Trenitalia che dall'esiguo residuo concesso al trasporto locale. All'articolo 25, infatti, viene istituito un fondo per gli investimenti del gruppo FS finalizzato alla conclusione dei nuovi contratti di servizio, ma si ignora totalmente una parte significativa del trasporto locale e cioè quello ferroviario. È del tutto incomprensibile come si possa immaginare una strategia di rilancio e potenziamento del trasporto ferroviario regionale se non vengono coinvolte le realtà delle ferrovie regionali e locali che, vorrei ricordare a tutti noi, servono 5.000 Comuni

Ogni giorno in Italia circa 15 milioni di persone utilizzano autobus, tram, metropolitane e traghetti. Se si pensa che i passeggeri di FS sono un milione e mezzo al giorno, è facile comprendere come il trasporto pubblico locale non sia solo uno dei servizi sui quali si misura la capacità di risposta delle Regioni e dei Comuni, ma un volano importante per l'economia del nostro Paese. Ma su questo punto il vostro decreto-legge anticrisi contraddice il vostro federalismo, svelando così una delle prime colossali bugie che avete raccontato al Paese. Il secondo punto sul quale mi voglio soffermare riguarda il sostegno alle imprese in questo momento di difficoltà di accesso al credito e di stretta finanziaria. Vi sono imprese sane che da mesi, talvolta anni, sono in attesa di vedersi riconosciuti dallo Stato i pagamenti a loro spettanti, pur avendo continuato a garantire agli utenti il regolare svolgimento dei servizi. Ciò condanna molte aziende sane ad una crisi pesante sul versante della continuità ad operare nel sistema economico, con la conseguente caduta verticale di buona parte dell'occupazione diretta e nelle attività dell'indotto. Questa Questa vostra undicesima richiesta di fiducia è un errore ed il rifiuto a ogni modifica migliorativa del decreto-legge in esame non potrà che produrre le contraddizioni e le difficoltà che abbiamo ripetutamente segnalato in questi mesi. però, purtroppo, è la vostra idea dell'Italia: non un grande Paese in grado di uscire con una politica solidale di alto profilo dalle attuali difficoltà sociali ed economiche, ma un'Italia piccola, ripiegata su se stessa ed incapace di affrontare a viso aperto il futuro del proprio destino. Per questo non meritate la fiducia di quella parte dell'elettorato che è ancora vasto ed attivo e che noi rappresentiamo, che non smette di sperare in un futuro migliore al quale voi, purtroppo, avete dimostrato di non voler appartenere.

vorrei cominciare il mio intervento ricordando ai pochi presenti in Aula le parole contenute nel messaggio di fine d'anno del Presidente della Repubblica, parole come sempre di saggezza, di equilibrio, come sempre osannate da tutti, maggioranza, opposizione, Governo, società civile. Il presidente Napolitano, dando così vera e costruttiva speranza al Paese - altro che il richiamo al vacuo ottimismo che ogni tanto fa il Presidente del Consiglio ci ha detto che dalla crisi economica, finanziaria e sociale che ha ormai investito anche l'Italia si può uscire meglio di come vi si è entrati. Ha usato questa bellissima espressione: «può uscire una società più giusta». E ci ha ricordato che per farlo è necessario cercare di assumere provvedimenti condivisi con le parti sociali e, se possibile, tra maggioranza e opposizione. Ma il Governo e la maggioranza si sono comportati in modo diametralmente opposto.

si possono superare gli steccati e i limiti ideologici e fare davvero l'interesse del Paese. Ma c'è di più e, anzi, di peggio. Questo provvedimento reca una dizione molto importante e molto significativa: «misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» ma, purtroppo, tra il titolo e i contenuti del provvedimento non vi è alcuna corrispondenza. Non siamo assolutamente in condizione di affrontare in un quadro strategico nazionale misure anticrisi per sostenere famiglie, lavoro ed imprese. sia importante sottolinearlo perché ci troviamo di fronte ad un Governo ed al suo Ministro dell'economia che per mesi ci hanno detto che tutto avevano capito e tutto avevano anticipato e che "avevano messo al riparo l'Italia dalle conseguenze di un'eventuale crisi". Invece, i risultati di alcuni provvedimenti sbandierati come panacea sono già negativi e sotto gli occhi di tutti, dall'abolizione dell'ICI alla detassazione degli straordinari: tutte misure che invece che sostenere o prevenire hanno comportato danni e più volte, come nel caso della Robin Hood *tax*, è stato necessario rivedere le decisioni e correre a tardivi ripari. Ma andiamo avanti. Un'Italia più giusta, auspicava il Presidente. Noi sappiamo che le cause della crisi economica sono da ricercare in gran parte fuori dal nostro Paese, ma sappiamo anche che essa colpisce i Paesi anche a secondo della loro capacità di reazione; colpisce i Paesi che sono in grado di reagire perché hanno gli strumenti per farlo ed altri che, invece, hanno più difficoltà. Quando pensiamo all'Italia pensiamo ad un Paese che presenta la più grande distanza tra le aree sviluppate e quelle meno sviluppate, una distanza che, come

Il Governo e la maggioranza non fanno davvero nulla per invertire questa drammatica tendenza, anzi, dall'inizio dell'attuale legislatura viene portata avanti una sistematica azione di svuotamento degli interventi di investimento produttivo nelle aree più deboli del Paese che sono tra le poche misure che bisognerebbe adottare per aggredire la crisi. Se la crisi è frutto di disuguaglianza la prima cosa da fare è proprio favorire lo sviluppo nelle zone deboli del Paese e contemporaneamente venire incontro, come diceva poc'anzi la collega Baio, ai ceti deboli del Paese. Ma se questo è vero, non si possono usare le risorse destinate alle zone deboli del Paese per fare tutto quello che si vuole, per mettere delle toppe. Non è possibile tagliare 16,600 miliardi di FAS, come è stato fatto finora, con la motivazione risibile che, siccome le amministrazioni di quelle aree, le classi dirigenti del Sud, non sono in grado di spendere i loro soldi, allora gli vengono tolti così si risolve il problema. Voglio ora fare due brevissime considerazioni. La prima non è mia ma del Presidente degli USA il quale, a chi gli chiedeva perché il Paese deve aiutare chi non ha saputo fare scelte oculate con i mutui, ha risposto: se il tuo vicino per una negligenza, per una cicca accesa, ha la sua casa che va a fuoco, tu pensi a spegnere l'incendio, anche perché sai che quello prima o poi si può allargare e colpire anche te e la tua casa. Se utilizziamo come spiegazione il fatto che il taglio è frutto dell'incapacità, condanniamo quelle aree, quei cittadini all'abbandono a vita e prima o poi quell'abbandono influenzerà anche il resto del Paese.

Perché questa consapevolezza non è un valore comune? Perché i nostri colleghi meridionali della maggioranza non si oppongono a ciò? Per esempio, al fatto che ancora una volta vengono penalizzate le aree del Sud con le imprese che dovranno pagare, grazie alla differenziazione delle tariffe energetiche, un costo maggiore? è un altro rischio spaventoso e, nel frattempo, sono stati cancellati tutti gli strumenti che avrebbero potuto portare più investimenti al Sud del Paese. Signora Presidente, allego al Resoconto il resto dell'intervento e concludo dicendo che proprio quell'Italia

Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, ancora una volta, per l'undicesima, malgrado vi sia una maggioranza consistente al Senato - 40 voti in più - e nonostante il comportamento limpido e trasparente dell'opposizione, che sia nelle Commissioni che in Aula non ha mai fatto il minimo accenno di ostruzionismo (addirittura neanche

Come altri senatori hanno già ricordato in quest'Aula, il combinato disposto decreto-legge voto di fiducia, in una condizione che vede questa maggioranza schiacciante, finisce per calpestare le prerogative parlamentari ed impedisce di apportare qualche miglioramento, che invece sarebbe doveroso e persino necessario a questo provvedimento anticrisi. Con il contributo dell'opposizione avevamo presentato alcuni emendamenti ed eravamo anche disponibili, in Commissione, a ridurli. Innanzitutto, si potevano tagliare gli sprechi e devolverli al sostegno duraturo dei salari, cioè ad una vera e propria redistribuzione del reddito; tassare i redditi miliardari e puntare sulla crescita e sulle nuove risorse tributarie che essa avrebbe determinato. Il *bonus* per le famiglie è la ripetizione dell'intervento effettuato dal Governo Prodi nel 2007, quando il PIL era intorno al 2 Nel 2007 il *bonus* aveva senso in quanto si perseguiva una finalità redistributiva. Oggi, date le condizioni attuali ed attese dell'economia, sarebbe stato necessario un intervento di portata ben più ampia, sia per importo medio che per numero di contribuenti interessati. Data la necessità di sostenere anche i redditi medi - anche il ceto medio soffrendo i morsi della crisi - la misura da attuare sarebbe stata un innalzamento permanente delle detrazioni per un importo medio almeno di 500 euro l'anno per i redditi da lavoro e da pensione. Abbiamo già parlato anche ieri dell'autorizzazione in bianco data all'utilizzo della Cassa depositi e prestiti, ossia ai risparmi dei vecchi, degli italiani. Infatti le Poste stanno anche dove non ci sono le banche, anche nei paesini sperduti. Si dà carta bianca al Ministro dell'economia nell'erogazione dei risparmi pubblici. Noi non siamo contrari a fare la concorrenza al settore bancario, per carità, perché la concorrenza è sempre amica dei consumatori e dei risparmiatori. Però, quando si concede questa carta in bianco al Ministro dell'economia senza la necessaria trasparenza, vuol dire dare un potere discrezionale, che può avere dei pericoli. Non abbiamo detto che tutto era da buttare di questa manovra. Avevamo detto che il *bonus* delle famiglie andava bene, il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, l'IVA da pagare al momento dell'incasso, gli sconti sull'IRES e sull'IRAP, il blocco delle tariffe ferroviarie in favore dei pendolari, la detassazione degli straordinari (che in tempi di recessione sembra quasi una beffa). Non va invece bene non aver detassato i salari e le pensioni. Il ministro Tremonti ha sempre parlato della necessità di evitare i benefici a pioggia e di concentrarli su pochissimi obiettivi, soprattutto in un periodo di penuria e di scarsità. Ha fatto invece esattamente il contrario ed è per questo che la sua non è una manovra, ma uno stillicidio di interventi disseminati in 36 articoli. Bastava concentrare tutte le risorse disponibili sulla detassazione dei salari al di sotto di una soglia di 30.000 euro di reddito. Non parliamo poi della ciliegina sulla torta, quella dell'IVA dal 10 al 20 per cento sui contratti di SKY, che si riverbererà su 4 milioni di famiglie. Ma quando non si ha la diretta percezione di una crisi che viene da lontano, che risale almeno al 7 agosto 2007, data del primo allarme dei *subprime*; quando si gioca con la «manovrina anticrisi» alla stessa stregua dei prestigiatori con il gioco delle tre carte, come ha giocato il ministro Tremonti,

(gli stessi soldi che sono stati sperperati per salvare i capitani coraggiosi, quelli di Alitalia); quando si promette di utilizzare fondi europei già assegnati alle Regioni, non si compiono quegli atti necessari di cui i precari, le famiglie, le imprese e i lavoratori avrebbero bisogno per approntare un piano straordinario di uscita dal tunnel della crisi.

Immaginiamo quei tributaristi mediocri quali danni faranno al Paese con manovre di puro stampo illusionistico e da commedia degli inganni.

*(PD)*. Signora Presidente, già altri colleghi, in maniera molto più autorevole di quanto non possa fare io, hanno segnalato l'assoluta incongruità tra

Pur considerando il limite dell'efficacia di un intervento in un'Aula praticamente deserta, a futura memoria forse sarà comunque il caso di segnalare la piena presa di coscienza, la piena consapevolezza che il nostro partito ha riguardo a questo ennesimo inganno.

ed assolutamente distratto, distante ed estraneo rispetto alle effettive necessità del Paese. Però questo decreto serve per fare cassa dal punto di vista dell'*audience*; serve per continuare questa commedia degli inganni; serve per continuare a far credere al popolo italiano che a a Roma c'è un Governo che governa e che decide, il cui Capo può tranquillamente anche permettersi il lusso di trascorrere tre o quattro giorni la settimana in Sardegna Ho parlato di paradossi. Ne vorrei sottolineare uno in maniera molto esplicita. I vari rappresentanti del Popolo della Libertà, della Lega e del Governo, quando vengono opportunamente interrogati riguardo all'effettiva efficacia di questo provvedimento a beneficio dei lavoratori dipendenti, all'unisono, come in un ritornello ormai stantio, dicono che in questo provvedimento c'è la detassazione degli straordinari. Questa è una beffa nella beffa, perché di straordinari in Italia non ne fa più nessuno. Questo è un Paese ormai allo sbando, un Paese in cui la cassa integrazione non basta più, tante sono le persone che ne hanno bisogno; è un Paese che, alla stessa stregua degli altri Paesi d'Europa, probabilmente dovrebbe interrogarsi su come organizzare meglio il lavoro ordinario, piuttosto che parlare di lavoro straordinario. C'è il problema della sopravvivenza, figuriamoci se possono essere attenuati i bisogni, ristorati i morsi della fame dei lavoratori dipendenti detassando un istituto, quello degli straordinari, che ormai è scomparso dal nostro Paese. Mi chiedo se ci sia un po' di malafede in questo provvedimento e se qualche burlone, solito a raccontare le barzellette nelle piazze d'Italia, abbia voluto inserire questo elemento per indurre all'ottimismo e magari costringere qualcuno anche ad aumentare il livello dei consumi con i soldi che non ha. Inoltre, a costo di essere ripetitivo, vorrei esprimere il mio personale parere riguardo a quella che considero la vergogna della *social card*. Checché se ne possa dire, checché si possa affermare che più che l'onor poté il digiuno, credo non sia lecito e consentito determinare pseudoprovvedimenti governativi mettendo in discussione e mortificando la dignità delle persone. La certificazione della propria indigenza costituisce la peggiore gogna che un Governo possa determinare a carico di quanti dovrebbero essere i più sostenuti, i più aiutati, per l'appunto i deboli. Questa misura è strutturalmente evanescente, politicamente e socialmente dannosa e pericolosa.

30.000 uomini appartenenti alle Forze armate che, come un sol uomo, verranno dispiegati e impiegati nel territorio italiano per risolvere tutti i problemi dell'ordine pubblico, stupri compresi. Credo che questo sia un esempio di schizofrenia che andrebbe esaminato proprio clinicamente, perché a tutto deve esserci un limite, non è possibile che basti avere lo stemma della Presidenza del Consiglio alle spalle per poter sparare le peggiori sciocchezze: 30.000 uomini presi dalle Forze armate rappresentano un inganno, una stupidità assoluta, sono la manifestazione più concreta di quanto siano di quanto siano poco chiare le idee di chi ci governa. Vorrei dare una risposta finale con gli ultimi secondi a il nostro Paese, che ha già cinque corpi di polizia, con l'immissione della Marina, dell'Aeronautica e dell'Esercito, avrebbe otto corpi di polizia e questo avverrebbe

Si dice che in Italia funzioni il bicameralismo perfetto, ma in realtà l'esperienza degli ultimi anni e soprattutto degli ultimi mesi mostra una smagliatura all'interno di questa impostazione.

in questo modo i termini classici del confronto tra i due rami del Parlamento vengono sostanzialmente vanificati. La vanificazione è tanto più evidente quando si vedono provvedimenti che hanno quasi esclusivamente la forma di decreto, con dubbi estremi su necessità, urgenza, premesse di costituzionalità e così via, che vengono affrontati con la massima rapidità e poi risolti quasi quasi istantaneamente con la fiducia. Dopodiché, l'idea che si possa discutere nell'altra Camera di una questione che è stata così contratta e risolta con la fiducia si perde, per cui nella Camera successiva il dibattito è ancora più contratto e

sul cosiddetto bicameralismo perfetto, sull'autonomia delle Assemblee elettive. Un giorno o l'altro, il Presidente del Consiglio dovrà decidersi a venire a trattare questo argomento in quest'Aula che solitamente diserta. di legge anticrisi, c'è un'evidente sproporzione tra la natura della crisi e i provvedimenti. appartiene in grandissima parte ad un contesto internazionale che è complicatissimo, su cui non entro, però ci sono degli aspetti specifici della crisi italica che vengono dimenticati. Dal mio punto di vista, dal punto di vista del Gruppo dell'Italia dei Valori, l'elemento fondamentale, che poi riunisce tutti gli altri, è la caduta del potere d'acquisto dei salari, delle pensioni e un sostanziale drastico peggioramento delle condizioni di vita che non può essere fatto dimenticare dalla tecnica mediatica in uso da qualche tempo, che cerca di persuadere gli impersuadibili

a come è stato gestito, malissimo, il cambio della moneta. Il centrodestra ha sempre fatto scandalo sulla questione dell'euro di Prodi sollevando un polverone pazzesco, ma in realtà il danno effettivo della gestione del cambio del cambio di moneta non dipende tanto da quello che il centrodestra ha sostenuto, cioè l'errata valutazione della lira in confronto all'euro, quanto dal fatto che l'assoluta mancanza di controlli, il liberismo più sfrenato dato a chi aveva il potere di utilizzarlo ha determinato una redistribuzione della ricchezza forzosa all'interno della società italiana. In tal modo, i redditi da lavoro si sono nettamente sono nettamente impoveriti e ci sono dei ceti, in parte chiaramente identificabili, in parte meno, un po' misteriosi, ma sostanzialmente i ceti dell'intermediazione, che sono riusciti a fare aggio sulla moneta e hanno trasformato il passaggio dalla lira all'euro in un'occasione di appropriazione privatistica di risorse economiche collettive. Il secondo elemento è una politica fiscale che il centrodestra ha sempre fatto nettamente, anche dichiaratamente, senza timore di preoccuparsi troppo, a vantaggio dei ricchi e degli evasori. Questo ha aggravato il male. Il terzo punto è più oscuro, è meno noto, però è importante anch'esso, ed è il fatto che costantemente i tassi d'inflazione programmata sono stati sempre regolarmente al di sotto dell'inflazione reale. C'è una sorta di lotta tra mondo ufficiale e mondo reale nell'economia che si combatte a tutto danno del mondo reale. quarto elemento, che strategicamente è il più disastroso nel futuro, è quello della diffusione con tutti i mezzi possibili e immaginabili del lavoro precario, che porta con sé una quantità di conseguenze di cui certamente alcune parti politiche possono essere soddisfatte. Per esempio, la diffusione estrema del lavoro precario comporta l'indebolimento dei sindacati. È evidente che nella situazione odierna ci sono parti politiche che possono gioire di questo fatto, ossia che il sindacato sia ridotto ormai sullo sfondo nella scena economica. I Ministri teorizzano che il conflitto del lavoro ormai non ha più ragione di esistere e la ragione e la ragione è molto semplice, perché il conflitto lo governano solo loro, direttamente, a vantaggio dei poteri economici. La manovra, nel complesso, è inesistente. Altri colleghi hanno già riferito alcune grandezze, però è interessante ricordarle, perché il Servizio bilancio della Camera, non un punto di vista di parte, ricorda che il piano di Tremonti

c'è addirittura un rovesciamento: invece di esservi un saldo passivo di impegno, c'è un saldo attivo di 390, e c'è chi dice anche 500 milioni. Il saldo positivo significa che invece di mettere risorse si levano, e quindi in realtà è una manovra in «levare», invece che in «mettere». Cosa si sarebbe dovuto fare? O aumentare la spesa pubblica o ridurre la pressione fiscale. Invece, l'incremento netto delle entrate previste funziona solo per compensare le spese e questo contrasta con la visione classica, comunemente accettata, per cui in recessione l'unica vera e autentica soluzione per risolvere i problemi è darsi da fare per far ripartire l'economia. Questa manovra non ha alcun carattere

nel quadro europeo ci saranno iniziative di stimolo fiscale in questa direzione, mentre in Italia questo tipo di impegno non ci sarà.

del Governo. Entro certi limiti, se il Governo fosse del tutto coerente con la sua impostazione gli si potrebbe riconoscere se non altro la virtù della fermezza. Invece, in realtà, c'è un Governo che sceglie una manovra che fa il solletico alla crisi economica, finge di affrontare i problemi sostanziali, risparmia, non tira fuori risorse, ma poi le dilapida in voragini vertiginose.

ci sono alcune dispersioni di fondi pubblici che sono veramente impressionanti: ricordo, signora Presidente, che sono stati sottratti ai Comuni circa 3miliardi, con l'abolizione dell'unica imposta federalista che c'era in questo Paese. Questa è una frase fatta, lo so: è già stata detta tante volte. Tuttavia, vale la pena di ripeterla, perché se c'era una possibilità per i Comuni di gestire una certa grandezza economica autonoma era quella; è stata tolta di mezzo e la ricompensa non è pari alla sottrazione. Poi c'è la dispersione dei fondi nell'Alitalia, che è impressionante: 4-5 miliardi che saranno pagati dai cittadini, perché si sono voluti togliere i debiti dall'impresa, insaccarli tutti dentro un'altra falsa impresa e permettere all'Alitalia di accedere poi ad una trattativa dinamica con i capitani coraggiosi. L'Air France, tra quattro anni, probabilmente potrà avere quasi gratis l'impresa che avrebbe pagato e di cui si sarebbe assunta

sia un fatto doveroso ed importante per questo Parlamento e per questo Governo. Vorrei però tornare al provvedimento in discussione: si è sentito dire che è insufficiente, limitato ed incompleto. I pregi sono

della propria finanza, del proprio debito pubblico complessivo non efficiente e non efficace con un saldo negativo, specialmente di parte corrente,

la ripresa ed una certezza di recupero dopo questo momento di crisi. Bisogna però anche riconoscere che, in tutti questi anni, non si è avuto il coraggio di affrontare una riforma importante e fondamentale del nostro Paese che riguardava, ad esempio, anche la finanza: si tratta del federalismo fiscale che, finalmente, sotto pressione, dopo molti anni di impegno e di costanza da parte della Lega, finalmente è arrivato in porto ed è stato positivamente evaso da questo ramo del Parlamento con un lavoro molto importante di approfondimento. In questo caso

che dà e deve dare fiducia alle imprese e far comprendere che vi sono dei primi interventi per la famiglia e per il sostegno delle persone svantaggiate, nonché segnali importanti per la ripresa economica, per le piccole e medie imprese, il vero tessuto portante del nostro Paese, in

fondamentale, che ormai è diventato patrimonio di tutti noi, dei costi standard, superando i costi storici e quindi superando definitivamente questo modello di crisi che ci ha visto, non dico impreparati, ma sicuramente deboli, perché in questi trent'anni forse siamo stati troppo leggeri nella nostra economia. PRESIDENTE.

con il decreto-legge n. 185 il Governo introduce un insieme di norme dirette a fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale, favorendo l'incremento del potere di acquisto delle famiglie, il sostegno al lavoro, all'occupazione ed alla competitività del Paese. Una manovra anticrisi che, nel complesso, tra spese ed entrate vale oltre 5,5 miliardi di euro, ma che non include al suo interno disposizioni esplicitamente riconducibili alla risoluzione della crisi che sta interessando il settore agroalimentare e della pesca né, tanto meno, misure specifiche per il suo rilancio competitivo. All'interno di un decreto-legge volto all'incentivazione delle imprese e dell'occupazione e che mira a «ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale» è inaccettabile dover constatare la totale assenza di interventi finalizzati al rilancio competitivo del settore agroalimentare. Ed è spiacevole anche considerare che in tutti i Paesi europei, dove si stanno affrontando decreti anticrisi,

Come già accaduto nel corso dei primi mesi di questa legislatura (ricordo il Documento di programmazione economico-finanziaria, il decreto-legge n. 112, ma anche la legge finanziaria), ancora una volta l'agroalimentare, e con esso le tante eccellenze del *made in Italy*, viene messo da parte da un Governo che, invece di dare ascolto alle segnalazioni sullo stato di crisi del comparto provenienti dal mondo produttivo e dai senatori del Gruppo del Partito Democratico in Commissione agricoltura, ha deciso di intervenire operando vistosi tagli. Un Governo che non intende assumersi la responsabilità di provvedere al sostegno ed al rilancio competitivo dell'agricoltura italiana che, invece, necessita urgentemente di un progetto strategico, che abbia una prospettiva di ampio respiro e che sappia attivare interventi strutturali profondi. Anche quando siamo riusciti in questa Aula, dopo innumerevoli sforzi, ad ottenere qualche modesto risultato, si è verificato che alla prima occasione utile il risultato conseguito sia stato ridimensionato dal Governo, quasi sempre a causa della riduzione dell'originaria copertura finanziaria. Mi riferisco, signora Presidente, al decreto-legge n. 207, cosiddetto proroga termini, dello scorso 30 dicembre, al cui interno il Ministro dell'economia ha previsto la soppressione e l'abrogazione di disposizioni a sostegno dell'agricoltura e della pesca approvate solo poche ore prima nella legge di conversione del decreto-legge n. 171, così come il collega Andria ha segnalato nel suo intervento di ieri. misure importanti che vengono a mancare in un momento in cui gli elementi di debolezza del comparto agroalimentare sono amplificati dalla volatilità dei prezzi, dalle inedite difficoltà di accesso al credito e da un ruolo sempre meno incisivo del sostegno pubblico. Un settore, quello dell'agricoltura e della pesca, signora Presidente, che come più volte ribadito dai banchi di quest'Aula sta attraversando una delle fasi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi e gli oneri sociali sono raddoppiati,

Di contro, i prezzi all'origine, dopo una fase di rialzo nella prima metà dello scorso anno, sono in caduta libera: stando agli ultimi dati disponibili, sono scesi in media del 7 con punte del 35-50 per cento per il mercato dei cereali. E in effetti, già lo stiamo vedendo sul livello dei redditi degli agricoltori, che dopo l'impennata del 2008 ovunque segnala un calo.

Una crisi testimoniata a gran voce da tutte le organizzazioni professionali e sindacali del settore che abbiamo ascoltato in Commissione agricoltura durante le numerose audizioni svolte nel corso degli ultimi mesi. Voglio però citare anche le manifestazioni di piazza che hanno interessato importanti organizzazioni agricole del nostro Paese. In tale contesto, attraverso gli emendamenti presentati dal Gruppo PD in Commissione agricoltura al disegno di legge in discussione, avevamo chiesto - anche se purtroppo, ancora una volta, inascoltati - di reperire le risorse necessarie ad attivare immediatamente una serie di misure straordinarie, richieste a gran voce da tutta la filiera, per rilanciare e sostenere il settore agroalimentare. Avevamo previsto il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, finanziato nelle precedenti leggi finanziarie, cui invece importanti risorse finanziarie sono state tolte da questo Governo.

dotazione del fondo istituito per le azioni a sostengo del *made in Italy*, prima da noi aumentato, anche con il plauso del Governo, poi eliminato nella legge successiva.

ieri i lavoratori della FIAT Auto di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, una realtà fino a poco tempo fa simbolo dell'industrializzazione nel nostro territorio, nel nostro territorio, sono stati qui a manifestare davanti a Palazzo Chigi. Gli operai, molti dei quali giovani e fortemente professionalizzati, sono esasperati dall'aver dovuto affrontare uno dei periodi più lunghi di cassa integrazione. Quella che è stata per decenni il fiore all'occhiello della produzione industriale del Sud d'Italia è oggi un luogo di preoccupazione e di incertezza. Da quella fabbrica sono state prodotte auto esportate in tutta Europa e in tutto il mondo. Ebbene, l'anno scorso a Pomigliano si è lavorato soltanto due mesi e, per quest'anno, la previsione è di qualche settimana in più. Ma non ci sono altre certezze. Gli oltre 5.000 lavoratori non hanno certezza sul proprio futuro. Non è soltanto una preoccupazione occupazionale, non è questo l'unico motivo che ci spinge ad intervenire. L'azienda finora non ha assegnato, né intende farlo, una nuova missione produttiva all'impresa di Pomigliano. Se questo non accadrà, ci sarà un ridimensionamento dello stabilimento e quindi dell'organico. Sottolineo che c'è un indotto che riguarda circa 30.000 persone stiamo parlando di una realtà in cui le famiglie sono generalmente monoreddito. In tal caso, quindi, verrebbe a mancare l'unico esiguo - più basso che in altre aree del Paese - reddito. Se questo reddito viene a mancare, è la disperazione. Temiamo che la crisi economica, tuttora sottovalutata, almeno nelle contromisure del Governo, come abbiamo detto finora, possa definitivamente piegare ogni capacità di ripresa di tante aree del Sud e in particolare delle zone produttive. Ci sono state iniziative da parte della Regione Campania, il cui presidente ha scritto al Presidente del Consiglio dei ministri, ma non c'è ancora alcuna risposta a tale grave questione.

risparmiatori, ai quali il Governo aveva promesso che non avrebbero perso un euro, non hanno più nulla: i titoli, le azioni e le obbligazioni Alitalia sono diventati carta straccia.

La cifra che riguarda questi ultimi è di circa 300 milioni di euro e, per quanto concerne gli azionisti, il valore derivante dall'ultima quotazione (0,445 euro ad azione) è pari ad oltre 600 milioni di euro. È dal 4 giugno 2008 che la Consob ha disposto la sospensione in via cautelativa e a tutela del mercato dei titoli Alitalia, per scongiurare i rischi di eventuali speculazioni. Da allora, decine di migliaia di risparmiatori che avevano in mano i titoli non solo non hanno più potuto negoziarli,

La seduta è tolta